con la normativa nazionale e comunitaria in materia di raccolta differenziata si inserisce in un più complesso quadro normativo. Quanto sancito con il predetto articolo 5, che pone l'obbligo per i Comuni della Regione Campania di avvalersi in via esclusiva per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei Consorzi di bacino *ex* legge regionale n. 10 del 1993, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della Protezione civile n. 2948 del 1999, si pone in linea con le disposizioni vigenti e ne costituisce un mero atto consequenziale. Infatti, com'è noto, al fine di incrementare gli obiettivi della raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente con il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con legge 27 gennaio 2006, n. 21, con quanto previsto dal citato articolo 5, si è provveduto ad attribuire ai Consorzi di bacino, identificati con legge regionale della Campania n. 10 del 1993, il compito di effettuare la raccolta differenziata degli imballaggi primari ed eventualmente della frazione organica dei rifiuti ingombranti, nonché della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. Tale principio è stato ulteriormente ribadito con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, il cui articolo 3 sancisce che, al fine di consentire l'ulteriore implementazione della raccolta differenziata, è autorizzato, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un contributo a favore dei Consorzi stessi. Premesso ciò, si precisa che quanto disciplinato con le citate ordinanze nn. 3529 e 3564, oltre a garantire i contratti per l'affidamento della raccolta dei rifiuti già stipulati, ha un ambito applicativo limitato. Infatti, la previsione di un'attribuzione del servizio in via esclusiva ai Consorzi di bacino è limitata alla sola raccolta differenziata, ovvero solo ad una parte dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, e l'efficacia temporale di quanto disposto nelle ordinanze è destinata ad esaurirsi con il venir meno dello stato di emergenza. Pertanto, il servizio della raccolta differenziata in proprio, da parte dei Comuni interessati, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3564 del 2007, presenta sicuri profili di compatibilità con la vigente normativa in materia. In particolare, la gestione in proprio da parte dei Comuni costituisce un *minus* anche rispetto ai cosiddetti affidamenti *in house*, ovvero svolti nell'ambito della propria organizzazione, la cui ammissibilità, sia pure in casi limitati e con modalità restrittive, è stata espressa in numerose e recenti sentenze della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato. Inoltre, il Testo unico in materia ambientale prevede il trasferimento della competenza dei Comuni agli Ambiti territoriali ottimali (ATO), la cui individuazione territoriale coincide generalmente con quella della Provincia, al fine di pervenire a modelli di gestione integrata ed unitaria del servizio dei rifiuti, da erogare in area vasta, conseguendo economie di scala. Sempre in tale ottica, l'articolo 4 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recita testualmente: «I Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge della Regione Campania 20 febbraio 1993, n. 10» e la recente legge della Regione Campania n. 4 del 2007 recepisce la normativa di settore, prevedendo che gli ATO, acquisiscano le competenze originariamente attribuite ai Comuni. Appare del tutto evidente che le competenze in materia di rifiuti, attualmente attribuite ai Comuni, sono da considerarsi motivate dal regime emergenziale vigente, dovuto al commissariamento del settore dei rifiuti e dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, mentre le misure adottate per mezzo delle citate ordinanze sono finalizzate alla predisposizione dei modelli gestionali conformi alla normativa vigente. In tal senso deve essere interpretata anche l'ordinanza commissariale n. 215 del 2 luglio 2007, che ha incaricato i sub-commissari, Presidenti delle Province campane, nei relativi ambiti provinciali di competenza, a predisporre un programma di iniziative volto ad attuare, a livello provinciale, forme di collaborazione e coordinamento tra i Consorzi di bacino. Sempre con la medesima ordinanza n. 215, è stato attribuito ai Consorzi il compito di individuare modelli gestionali ed organizzativi del servizio dei rifiuti, in ambito consortile, provvedendo alla definizione della qualità del servizio e del cronoprogramma degli investimenti e degli interventi necessari al graduale raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, attraverso l'elaborazione di uno specifico piano industriale. Sulla base di tale programma, i Consorzi devono provvedere ad assicurare un servizio di raccolta differenziata secondo delle precise modalità, individuate nell'ordinanza stessa, come ad esempio la scelta di procedure di raccolta adeguate alle particolari caratteristiche del territorio. Si ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3564 siano in linea con le previsioni della normativa di settore, sia nazionale che regionale e, in particolare, con la recente legge regionale dei rifiuti n. 4 del 2007, che prevede il trasferimento delle competenze dei Consorzi di bacino ai futuri Ambiti territoriali ottimali. In relazione alla volontà dei Sindaci dei Comuni interessati di costituirsi in giudizio, si fa presente che i Comuni di Montecorvino Pugliano, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, San Mango Piemonte e Mercato San Severino hanno proposto ricorso TAR Lazio avverso l'ordinanza n. 3564 del 9 febbraio 2007. Il TAR, in data 9 maggio 2007, ha respinto le domande incidentali di sospensione dei Comuni.

raccolta differenziata l'affidamento esclusivo ai Consorzi costituiti con legge della Regione Campania n. 10 del 1993, e nella ulteriore considerazione che tale servizio prevede l'utilizzazione dei lavoratori assunti *ex* ordinanza ministeriale n. 2948 del 25 febbraio 1999. Tale favorevole assunto ha trovato conferma nella ordinanza del Consiglio di Stato n. 2106 del 2007 con la quale, in relazione ad analogo ricorso proposto dalla società General Enterprise, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittimo l'affidamento da parte del Comune di Vibonati ai consorzi di bacino del servizio di raccolta differenziata ordinando, per converso, al Comune medesimo di bandire una gara solo per l'affidamento della raccolta indifferenziata.

innanzi tutto ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la puntuale risposta, che però giunge un po' tardiva poiché la materia posta a oggetto dell'interrogazione del lontano 19 aprile è stata in parte superata dalla conversione in legge del decreto-legge

In realtà, la risposta è molto formale e puntuale, ma non soddisfa appieno tutte le perplessità che erano poste a base dell'interrogazione. La situazione della raccolta dei rifiuti in Campania era ed è ancora drammatica. L'interrogazione contestava l'obbligatorietà

si può mortificare i Comuni più efficienti (alcuni dei quali, direi la quasi maggioranza, si trovano in provincia di Salerno) che hanno raggiunto livelli di raccolta differenziata

con uno stipendio certamente non elevato, anzi forse insufficiente, per non far nulla, per non fare raccolta. Le immagini televisive sono sotto gli occhi anche dell'onorevole sottosegretario Naccarato, quindi concludo l'intervento dicendo che mi dichiaro soddisfatto per la parte formale e ovviamente insoddisfatto per la parte sostanziale, nonché preoccupato

vedrà nei prossimi mesi probabilmente esiti nuovamente sconvolgenti per noi, per il sistema Paese e disgraziatamente anche per l'immagine dell'Italia nel mondo.

Come correttamente riportato dall'onorevole interpellante, il TAR del Lazio, con sentenza n. 13559 del 2005, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2004, con il quale erano stati nominati i 29 membri di nomina governativa del CGIE. A seguito di questa sentenza, il Ministero degli affari esteri ha provveduto a riavviare, secondo le indicazioni elaborate dal TAR, le procedure previste per la nomina dei membri del CGIE limitatamente ai nove rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei patronati. In particolare, l'amministrazione ha aperto la procedura a tutti i sindacati e a tutti i patronati, inviando formale comunicazione a firma del vice ministro Danieli in data 22 giugno 2006. Tale comunicazione è stata inviata anche alle parti ricorrenti, specificando i criteri utilizzati per la selezione. Nel frattempo, il Ministero degli affari esteri aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio ed è in attesa della pronuncia sul merito da parte del superiore organo della giustizia amministrativa. Nella formulazione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati utilizzati gli elenchi dei patronati e delle organizzazioni sindacali e le indicazioni fornite dal competente Ministero del lavoro. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, sulla base delle indicazioni fatte pervenire dal Ministero del lavoro, la comunicazione indirizzata dal vice ministro Danieli alle organizzazioni sindacali precisava che «per la verifica del criterio di rappresentatività si terranno in considerazione i dati ufficiali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, basati sui seguenti elementi: consistenza numerica degli associati, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, formazione e stipulazione dei contratti nazionali del lavoro». Per quanto riguarda i patronati, invece, sono stati utilizzati i dati resi noti dal Ministero del lavoro attraverso la ripartizione del fondo patronati 2003, data dell'ultima rilevazione disponibile. Nella comunicazione inviata ai patronati è stato pertanto precisato che «la procedura di nomina prevede che la scelta venga effettuata esclusivamente tra gli enti che presentano in criteri previsti all'articolo 4, comma 5, della legge n. 389 del 1998. Si precisa, al riguardo, che per la verifica di tali criteri si terranno in considerazione i dati ufficiali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale». Trascorsi i 30 giorni previsti dall'articolo 5, comma 1, del regolamento, il Ministero degli affari esteri ha provveduto ad avviare le selezioni tra gli enti che hanno risposto alla comunicazione citata, sulla base dei criteri sopra enunciati. L'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ha così firmato un nuovo decreto di nomina dei 29 membri del CGIE, in data 7 settembre 2006, che è stato nuovamente impugnato dal CNA-EPASA, originando la sentenza del TAR del Lazio del 7 marzo 2007 che accoglie il ricorso. Questa amministrazione si è immediatamente conformata alla pronuncia del TAR, escludendo dalle attività del CGIE i nove rappresentanti delle Confederazioni oggetto del ricorso, ritenendo tuttavia che il Consiglio stesso fosse abilitato a continuare la sua attività, mentre nel contempo la Presidenza Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato anche contro la seconda sentenza, richiedendo di sospendere l'efficacia della sentenza del TAR del Lazio, in attesa di una pronuncia definitiva sul merito dell'intera questione. Tale richiesta è stata favorevolmente accolta dal Consiglio di Stato con l'ordinanza 3563 del 10 luglio 2007, che ha ritenuto fondati gli elementi presentati dal Governo. Pertanto, il CGIE può continuare ad operare legittimamente nella sua compagine normale di 94 membri, fintanto che non sarà intervenuta la pronuncia di merito del Consiglio di Stato su ambedue i ricorsi sopra menzionati.

i dati posseduti dal Ministero del lavoro circa la rappresentatività di questi patronati, di queste associazioni e di queste rappresentanze, anche se gli stessi sono fermi al 2003. Qui parliamo, però, di un organismo che deve rappresentare, l'appunto, gli interessi dei lavoratori, dipendenti e autonomi, e degli imprenditori che sono all'estero. Pur avendo grande considerazione e rispetto la Coldiretti, che in questo caso è stata privilegiata con un suo rappresentante in questo importante organismo, debbo rilevare che essa non possiede alcuna sede di rappresentanza all'estero, nè alcun patronato operante in nessuna Nazione

colgo però l'occasione per rappresentare all'onorevole Vice ministro l'importanza di valutare se in questo organismo debba essere privilegiata la rappresentanza di chi è più forte in Italia

di aprire un squarcio sulla questione aeroporti in Italia. Dopo anni di caos totale, il Ministero dei trasporti, non solo attraverso il Piano generale del trasporto aereo, ma anche attraverso il riordino e la possibilità di dare concessioni con le linee guida agli aeroporti con traffico inferiore ai 250.000 passeggeri,

al punto che gli enti pubblici sono dovuti intervenire destinando risorse che provengono sempre dai contribuenti. Per rimanere nell'ambito dell'interrogazione, che si riferisce all'aeroporto di Salerno-Pontecagnano, lo stesso è aperto al traffico civile ed è affidato in gestione parziale, a titolo precario, alla Società Aeroporto Salerno S.p.A, i cui azionisti, in base ai dati di bilancio dell'anno 2005, sono la Società Salerno Interporto S.p.A. (9 per cento) e il Consorzio Aeroporto Salerno (91 per cento). Dal 2006, l'ENAC ha avviato l'istruttoria relativa all'affidamento in concessione della gestione totale, *ex* regolamento n. 521 del 1997, all'esito della quale sarà possibile procedere alla sottoscrizione della convenzione regolante l'affidamento in gestione totale e alla approvazione ministeriale, con la predisposizione di un decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. In applicazione del decreto ministeriale n. 521 del 1997 e della circolare n. 12479 AC/1999, l'Ente ha rappresentato la sostanziale inapplicabilità dello stesso per aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri, passeggeri, nella media degli ultimi due anni o interessati da sola aviazione generale, dovuta a difficoltà tecniche in relazione alla consistenza delle previsioni di traffico e dei relativi piani di investimento, nonché dei piani economico-finanziari. Si è proceduto, pertanto, d'intesa con l'ENAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze, alla predisposizione di un apposito schema di direttiva, per la definizione di aggiornati criteri tecnico-economici, individuati sulla base del citato regolamento n. 521 Sinteticamente, sulla base di detta direttiva i soggetti titolari di gestione parziale aeroportuale, anche in regime di precariato (che hanno presentato istanza, ai sensi del decreto ministeriale per la concessione della gestione totale di aeroporti interessati da un traffico fino a 250.000 passeggeri e con possibilità di espansione, determinato sulla base della media accertata nell'ultimo biennio, o dalla sola aviazione generale), possono presentare all'ENAC un programma di intervento, comprensivo del piano degli investimenti e del piano economico-fìnanziario, elaborati secondo princìpi di prudenza con riferimento agli schemi stabiliti nella circolare ministeriale del 20 ottobre 1999, tenendo conto della consolidata scarsa movimentazione e dell'alta sensibilità a fenomeni estemporanei. L'ENAC, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti, senza ulteriori oneri per lo Stato, accerta preliminarmente il possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti previsti dal decreto ministeriale n. 521 del 1997 e l'avvenuto ripianamento delle perdite conseguite nell'ultimo bilancio di esercizio. L'istruttoria condotta sui programmi d'intervento è intesa a verifìcare che: gli investimenti previsti assicurino il mantenimento in operatività e sicurezza dell'aeroporto e siano coerenti con la caratterizzazione funzionale e la vocazione territoriale dell'aeroporto stesso; il piano economico-finanziario, tendente all'equilibrio, persegua obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione, evidenziando il possesso da parte delle società, sino al raggiungimento del predetto equilibrio, di un patrimonio netto atto ad assicurare, oltre al capitale sociale previsto dalle vigenti disposizioni, un adeguato apporto delle fonti di finanziamento necessarie a garantire l'attuazione degli investimenti previsti. Ciò al fine di evitare, come si diceva in premessa, il proliferare di aeroporti spesso a gestione fallimentare. Con il decreto di affidamento predisposto di concerto con gli altri Ministri interessati, viene determinato il periodo di durata della concessione, rilasciata fino ad un massimo di venti anni, in relazione alle valutazioni formulate con riferimento al programma di intervento ed alla tipologia dell'aeroporto. La durata della concessione è soggetta a revisione quadriennale in relazione all'attuazione del programma di intervento, con particolare riferimento alla realizzazione del piano degli investimenti e al raggiungimento degli obiettivi di "efficientamento". La direttiva n. 135/T del 12 settembre 2007 è stata controfirmata dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è attualmente al vaglio dell'organo di controllo per questioni formali di rito. In base ai dati attuali di traffico, l'aeroporto di Salerno rientra nell'ambito applicativo della suddetta direttiva con evidente possibilità di espansione del traffico commerciale, sia cargo che passeggeri, che lo stesso è in grado di attrarre. La società di gestione aeroportuale dello scalo in questione ha presentato la domanda con allegata una prima versione del programma di interventi sviluppato su un arco temporale di venti anni. Nel programma viene descritta ed analizzata l'attuale dotazione infrastrutturale, che negli ultimi anni è stata potenziata con la realizzazione di alcuni interventi, per un totale di circa 12 milioni di euro finanziati con risorse nazionali e regionali, di cui i principali sono: riqualifica della pavimentazione e prolungamento della pista di volo; regolarizzazione della RESA; strada perimetrale di servizio ed ispezione; riqualifica ed ampliamento del piazzale di sosta aeromobili; nuova aerostazione passeggeri;

prolungamento della pista di volo da 1.653 metri a 2.020 metri (sono in corso da parte della società di gestione le attività propedeutiche necessarie all'ampliamento del sedime);

Gli interventi in corso di realizzazione, attualmente in fase di ultimazione, e quelli programmati presuppongono, tuttavia, la disponibilità dell'intero sedime aeroportuale, compresa la quota parte del demanio militare. Si evidenzia che la disponibilità di tali aree potrà garantire il processo di sviluppo dell'aeroporto, dando valenza agli investimenti già realizzati e a quelli destinati a tale fine dal Governo nazionale e dalla Regione. In relazione allo stato di avanzamento dei lavori e all'andamento delle attività di certificazione dell'aeroporto, è prevista l'apertura dello stesso al traffico commerciale, merci e cargo, entro la fine del corrente anno.

Enti interessati: sulla reale operatività futura dello scalo in termini di voli giornalieri con le principali città italiane e dei Paesi confinanti e/o limitrofi;

I tecnici e il territorio danno previsioni ottimistiche sulla possibilità di intercettare i milioni di turisti,

metri», sono in corso, almeno per quanto ci dice la società di gestione, attività per concludere questa fase.

In realtà, non sono soddisfatto della risposta complessiva proprio perché conosco la vicenda di questo aeroporto in quanto, come ha ricordato l'onorevole Sottosegretario, ne ho fatto parte, anche se solo per qualche anno, nella qualità di componente del consiglio d'amministrazione, e le mie forti perplessità esistevano già allora e, malauguratamente, devo confermare che esistono Infatti, quell'aeroporto sconta una serie infinita di amministrazioni locali di centro-sinistra, compresa quelle provinciale e regionale, che hanno illuso, per decenni, il territorio di poter competere con l'aeroporto di Napoli-Capodichino e di poter prendere finalmente l'aereo

della concreta possibilità di aprire a voli di linea giornalieri. Tutto ciò non è stato reso possibile da una miope amministrazione politica che - sottolineo - è di centro‑sinistra, la quale non ha considerato il discorso della viabilità che è strettamente legata all'apertura di un aeroporto. Rammento

della viabilità, dei collegamenti, della metropolitana che non esiste e quant'altro, ma vi è anche un discorso urbanistico perché le amministrazioni dei vari Comuni interessati (Pontecagnano, Bellizzi e gli altri) hanno consentito di costruire in prossimità dell'aeroporto per cui ho serie preoccupazioni per l'agibilità dello stesso. sede, poi, rimarco la terza risposta, a mio avviso mancata, dell'onorevole Sottosegretario relativamente all'allungamento della pista. Penso che tutti quanti sappiano che non si può parlare di allungamento della pista ma di un suo completo rifacimento,

Questa, a mio personale avviso, è un'altra favola che viene propinata al territorio, che invece vorrebbe finalmente poter acquistare un biglietto d'aereo e poter partire da quell'aeroporto perché la richiesta

per amore di polemica) che questo aeroporto ha ricevuto tantissime visite di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari. Ebbene, spero che tutto questo, per lo meno per quelli che l'hanno visitato ultimamente, dia qualche concreto segnale di soluzione del problema perché alla base dell'interrogazione c'era proprio il fatto che, mentre il sottosegretario Annunziata,

ragione, e il giorno dopo quelle del suo Ministro che affermano l'esatto contrario, cioè che lui non vede prospettive, ecco forse questa sarebbe stata la risposta che avrei gradito di più. Grazie comunque.

con riferimento all'interrogazione in discussione faccio presente, in via preliminare, che riguardo al finanziamento degli istituti di patronato, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 7, della legge n. 152 del 2001, si applicano, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della medesima legge, i criteri di ripartizione del fondo patronati individuati dal decreto del Ministro del lavoro del 13 dicembre 1994, Tutti gli istituti in questione sono stati oggetto di visita ispettiva al fine di accertare, secondo le prescrizioni di legge, il loro grado organizzativo e di funzionalità, nonché l'attività svolta, adempimenti, questi, preliminari al fine della definitiva ripartizione dalle risorse finanziarie affluite al fondo patronati. In mancanza degli stessi non si può procedere, infatti, all'emanazione del decreto di ripartizione dei contributi affluiti al fondo patronati. Per quanto riguarda le verifiche ispettive relative all'attività 2004, oggetto specifico del presente atto ispettivo, sono in grado di informare che l'ultima relazione in merito è pervenuta agli uffici competenti nel mese di gennaio 2007. Nello stesso mese si è provveduto, quindi, ad elaborare il saldo definitivo, ai fini della stesura del successivo decreto interministeriale (Ministero del lavoro e dell'economia e delle finanze, firmato il 26 giugno scorso), con il quale si è provveduto alla ripartizione definitiva. I relativi ordinativi di pagamento sono stati inviati all'Ufficio centrale del bilancio il 18 luglio 2007 e da questo trasmessi, per via telematica, alla Banca d'Italia in data 27 luglio 2007. Colgo l'occasione, infine, per comunicare che il Ministero del lavoro intende emanare, in tempi brevi, il regolamento di cui all'articolo 13 della legge

Non si capisce per quale motivo non si possano modernizzare i metodi di controllo e di verifica. I patronati adesso sono in contatto e lavorano molto con l'INPS per via telematica, per quale motivo il lavoro ispettivo sui patronati sia rimasto indietro quanto alle modalità, cosa che crea ritardi e disagi notevoli ai patronati